Il presidente della 9[a] Commissione permanente, senatore De Carlo, riferisce sui lavori delle Commissioni riunite 8[a] e 9[a

Prendiamo atto del lavoro in corso, che mi pare sia arrivato a buon punto, visto che tre quarti degli articoli sono stati esaminati, salvo gli accantonati.

al valico di frontiera di Allenby, e che da un mese è in stato di arresto, con il timore che ci possa essere un processo arbitrario, in questo momento senza nessun capo di accusa. Dal momento dell’arresto risulta che si siano svolte quattro udienze, nelle quali

L’ultima delle quattro udienze si è svolta il 21 settembre e ha prorogato la custodia cautelare fino al primo ottobre, giorno nel quale si deciderà se far iniziare un processo penale. In quel caso però ci si attende che vengano formulate delle accuse. Questa mattina la moglie e il legale della famiglia hanno chiesto un pronunciamento del Governo italiano e una presa di posizione, ricordando evidentemente che Khaled è un cittadino italiano oltre che palestinese. Il legale Rossi Albertini ha avvertito che questa detenzione potrebbe tramutarsi in un vero e proprio processo penale, ma questa decisione sarebbe fondata su interrogatori viziati a monte dal fatto di di non essere stati resi in presenza di un difensore. Secondo il legale le autorità israeliane non hanno elementi per processarlo e, in ogni caso, si chiede al Governo di intervenire a tutela della libertà e dei diritti di un proprio cittadino.